«Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2009 quanto a euro 500.000 l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno 2010, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento del Ministero dell'interno e, per l'anno 2011, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

Colleghi, in attesa che la 5a Commissione permanente completi la stesura del parere reso sui residui emendamenti, sospendo la seduta sino alle ore 17.

Signor Presidente, ieri pomeriggio, in sua assenza, si è verificato più volte un episodio spiacevole che - ahinoi! - continua a caratterizzare alcune fasi del nostro lavoro in Aula, quando

prevede l'obbligo, per chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile, di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 10.0.3000, 32-*bis*.0.301, 32-*bis*.0.302, 32-*bis*.0.303, 32-*bis*.0.304 e 33-*decies*.0.300, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 32-*bis*.0.301 e 32-*bis*.0.302. Esprime poi parere di semplice contrarietà sulla proposta 33-*decies*.0.300, Esprime, infine, parere di semplice contrarietà sulla proposta 32-*bis*.0.303, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 2 le parole: "di cui al comma 3" siano sostituite dalle altre: "di cui ai commi 3 e 4" e che sia aggiunto poi il seguente comma: "3-*bis*. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società Poste Italiane spa nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole al prenditore, nel presupposto che l'emendamento

finestra"). Colleghi, informo che nelle nostre tribune sono presenti gli alunni dell'istituto «Santa Maria degli Angeli Madri Orsoline» di Brescia, che salutiamo.

una palese estraneità alla materia: abbiamo discusso di energia nucleare e di sostegno alle imprese e davvero non si capisce come si possa infilare in questo provvedimento anche una quella che interessa i servizi ferroviari. Si parla di liberalizzazione, di nuove norme per i contratti delle ferrovie regionali, si parla di servizio universale.

Grazie, Abbiamo conferito alle reti di impresa, che sono un'entità nuova e che tutte le volte si dovrà identificare in forma nuova,

ha posto delle riserve, gli stessi trattamenti di vantaggio fiscale dei distretti industriali. Noi voteremo a favore di tale emendamento e vorremmo anche chiedere un ordine del giorno del Senato

all'interno di un distretto, ovverosia alle imprese che si collegano sul territorio per migliorare il loro prodotto e per l'innovazione, una serie di agevolazioni che possono portare il sistema delle imprese a un salto in avanti, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

intende introdurre, infatti, è molto ampia e complessa e riguarda questioni sia di diritto sostanziale penale, cioè le modifiche in tema di reati di contraffazione, alterazione, o uso di marchi segni distintivi, brevetti, modelli e disegni, per i quali si prevedono pene più gravi e specifiche, sia di natura processuale che concernono la confisca obbligatoria, la competenza della procura distrettuale e la materia penitenziaria.

della competenza alla procura distrettuale anche per i reati in materia di contraffazione, alterazione o uso di marchi, collegati

Faccio presente che se si tratta di associazione per delinquere aggravata dallo stampo mafioso in senso lato è competente la procura distrettuale, tutte le altre associazioni per delinquere che possiamo definire semplici rientrano nella competenza della procura ordinaria. Estendere questo sistema ed attribuire competenze per reati

di doversi occupare di una infinità di reati che poco hanno a che fare con le competenze specifiche in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso. D'altra parte, se di fatto dovessero emergere elementi a sostegno dell'accusa di criminalità organizzata,

vorrei che avessero una sorte diversa le obiezioni che avanziamo sull'articolo 9. L'avevamo accantonato perché sembrava inopportuno accentrare ulteriormente sulla procura della Repubblica del capoluogo di distretto

tanto che il senatore Maritati è costretto anche in questa sede a presentare un ordine del giorno in cui supplica di incrementare le dotazioni organiche sui tribunali capoluogo di distretto, perché si stanno accumulando di volta in volta, in ogni riforma e in ogni testo, nuove competenze. Voglio precisare per i più distratti

Stiamo accentrando in maniera abnorme e disfunzionale indagini che non meritano di essere accentrate sul capoluogo di distretto. Siccome ciò non viola l'impianto del provvedimento ‑ mi rivolgo al Governo ‑ e non ne altera la sua natura

In Italia, i reati di contraffazione di marchio sono la grande maggioranza e incidono moltissimo sui marchi di altissima qualità della nostra produzione e anche sulle produzioni di nicchia di alta qualità delle piccole e piccolissime imprese. Pur tuttavia, non comprendendo perché vi sia questa differenziazione, le pene pecuniarie si alzano comunque rispetto alla situazione attuale. Siccome nella nostra intenzione si

perché qui si continuano ad attribuire competenze oltre misura alle procure distrettuali e con quest'ordine del giorno, di cui si è ampiamente discusso anche in Commissione, si chiede semplicemente lo stanziamento di adeguate risorse per quanto riguarda gli organici delle procure distrettuali in materia di criminalità organizzata. Esprimere parere contrario quando si chiede semplicemente di aumentare le risorse per svolgere le indagini in materia di criminalità mafiosa, camorristica e comunque organizzata mi sembra veramente un assurdo.

Dopo una consultazione non soltanto con i colleghi della Commissione bilancio, ma anche con colleghi che conoscono il merito della questione, naturalmente sulla base di una cognizione sommaria, posso esprimere parere di nulla osta

all'unanimità: «L'assenso del proponente, necessario all'aggiunta di firma ad emendamenti, è normalmente presunto, salvo tempestivo espresso diniego. In caso di ritiro da parte del proponente, gli altri firmatari possono mantenere l'emendamento, in conformità della disposizione di cui all'articolo 102, comma 6, del Regolamento, che consente a tutti i senatori di far propri gli emendamenti ritirati». approvata a maggioranza la seguente parte: «Conformemente alla prassi, quando il proponente ritira un emendamento per trasformarlo in ordine del giorno ai sensi dell'articolo 95, comma 7, del Regolamento, gli altri firmatari non possono chiedere la votazione dell'emendamento».

il primo firmatario chiede di trasformarlo in ordine del giorno, a quel punto che cosa avviene?

chiedere un impegno formale in quest'Aula, anche se non si è potuto formalizzare un ordine del giorno, affinché si possa, con provvedimenti o con misure che il Governo riterrà di adottare, salvaguardare la produzione artigianale e industriale italiana e garantire la necessaria trasparenza relativamente al ciclo di manifattura di un prodotto. Crediamo che la tutela e la valorizzazione del *made in Italy* siano

che possono finalmente farci assumere una posizione, coerente verso le nostre imprese e le nostre produzioni, di tutela dell'italianità delle produzioni

Adesso che il ciclo è ormai diventato cosmico, le produzioni italiane hanno un valore particolare che noi dobbiamo tutelare. [DE

il Governo è impegnato, ancor più alla luce di questo mandato parlamentare che condivide pienamente, su due fronti: affinché il Consiglio d'Europa adotti finalmente il regolamento già predisposto dalla Commissione europea su iniziativa italiana per rendere obbligatoria l'etichettatura con l'indicazione l'indicazione del Paese di origine su tutti i prodotti importati nell'Unione europea, e, nel contempo, sul fronte nazionale, come chiedono i proponenti, affinché sia valorizzata al massimo la produzione nazionale attraverso una maggiore riconoscibilità, e quindi attraverso un'eventuale tracciabilità della lavorazione dei singoli prodotti che vengono poi distribuiti sul territorio nazionale. Crediamo che questo debba essere un impegno comune del Governo e del Parlamento

Signor Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, collegato che siamo chiamati oggi ad approvare in quest'Aula risulta profondamente modificato nel suo complesso *iter* tanto da essere diventato un contenitore di eterogenee disposizioni che nulla o poco hanno a che fare tra loro, come per esempio le norme relative allo svolgimento del servizio ferroviario passeggeri in ambito nazionale e quelle in materia di servizio universale nonché di trasporto pubblico locale. Tuttavia, esso appare particolarmente urgente alla luce della forte crisi economica che ha investito e tuttora investe il nostro Paese e l'intera economia mondiale. Sono proprio le famiglie e le piccole imprese, vero collante del nostro tessuto sociale e produttivo, ad attraversare momenti difficili. Purtroppo, ancora una volta, il Governo, con il provvedimento in esame, ha perso una grande occasione per andare loro in soccorso formulando risposte adeguate e significative alle loro esigenze. In riferimento alla crisi economica, infatti, dalla presentazione del provvedimento ad oggi, molta acqua è passata sotto i ponti e il Governo sembra non essersene accorto. Le piccole e medie imprese, vera spina dorsale del nostro sistema produttivo, continuano a non aver quell'attenzione in termini di risorse, che meritano in un momento in cui sembrano essere le più esposte ai venti di crisi. In riferimento al provvedimento in esame ci preoccupano in particolare le modalità con cui si vogliono reindirizzare reindirizzare gli interventi per le aree sottoutilìzzate, rimodulare gli interventi inerenti i patti territoriali, la contrattazione negoziata e quindi gli accordi di programma. La disciplina di riordino degli strumenti di incentivazione e di aiuto alle imprese inciderà sulle risorse, in particolare sui FAS, e anche sulle competenze regionali in materia. Tale operazione sarà, tra l'altro, affidata ad una generica delega e non ad un coordinato meccanismo di norme di pronta applicazione. Troppo frequentemente in questo provvedimento si ricorre allo strumento della delega. Noi non siamo contrari per principio alle deleghe, tuttavia non le condividiamo quando, come nel caso in esame, difettano di princìpi direttivi e di criteri univoci tali da mettere il Parlamento nelle condizioni di non poter esprimere un parere articolato sui progetti di decreti legislativi. Non si può inoltre condividere la scelta di operare una rilevante riforma dell'azione collettiva risarcitoria rispetto alla quale associazioni di consumatori e numerosi cittadini rimasti vittime hanno assunto una posizione nettamente contraria non condividendo l'impostazione formulata dal Governo. Se ne altera lo spirito trasformandolo da strumento collettivo ad atto individuale cui poter aderire. Ma, in particolare, ci pare irragionevole disporne l'irretroattività e restringerne la portata alle posizioni "identiche" piuttosto che a "diritti ed interessi omogenei". Ci preoccupa inoltre la previsione di una sanzione al consumatore nel caso in cui non gli sia riconosciuta la *class action*. In tal modo il Governo sembra voler voltare le spalle alle migliaia di cittadini vittime dei grandi scandali finanziari che hanno segnato in modo così negativo l'economia italiana degli ultimi anni. Non appare inoltre condivisibile la scelta di concentrare presso il TAR del Lazio tutte le controversie attinenti alle procedure ed ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati in materia energetica. Con lo stesso ritardo con cui si prende atto dell'urgenza di sostenere l'impresa, in particolare nei suoi processi di internazionalizzazione, si tenta di avviare una nuova politica in materia energetica. L'Italia soffre

dal catastrofismo ideologico; siamo convinti piuttosto di avere un obbligo morale nei confronti delle future generazioni: quello di dover lasciar loro un pianeta non dico in condizioni migliori, ma almeno nelle stesse condizioni nelle quali lo abbiamo trovato. Per questo riteniamo quanto mai urgente promuovere e sviluppare le energie rinnovabili ed il nucleare, *in primis*, come ho detto, per ridurre la nostra dipendenza energetica dagli altri Paesi, ai fini di ridimensionare i costi dell'energia per le nostre imprese e per le nostre famiglie, mai come ora strangolate dalle difficoltà economiche. Colgo l'occasione per sollecitare nuovamente il Governo a semplificare le norme relative alla costruzione di centrali idroelettriche pubbliche nei parchi nazionali, trattandosi di un'energia pienamente rispettosa dei criteri criteri ambientali. Ad esempio, nel Parco nazionale dello Stelvio, dove l'abbondanza dell'acqua rappresenta un enorme potenziale di energia pulita pulita non sfruttata, la costruzione di suddette centrali potrebbe contribuire a ridurre ulteriormente la dipendenza energetica. Dobbiamo inoltre promuovere una cultura ambientale che parta dal risparmio energetico, anche in edilizia. A questo proposito mi riferisco al fatto che sarebbe opportuno prevedere nella progettazione di edifici pubblici il rispetto delle nuove tecnologie tecnologie volte al risparmio energetico, come già è stato fatto con successo nella Provincia di Bolzano con le cosiddette case clima. dell'efficienza energetica dobbiamo lavorare tantissimo, ancora di più, se consideriamo che questo è uno dei settori nei quali il nostro Paese è rimasto più indietro. Il ritardo non è tanto imputabile al privato quanto ai Governi, che hanno fatto ben poco fino ad ora, al contrario che in altri Paesi. Vi è dunque bisogno di dare segnali nuovi, a partire innanzi tutto dal sostegno alla ricerca, all'utilizzo delle nuove tecnologie, all'infrastrutturazione energetica. Il Governo su tali tematiche si è dimostrato disponibile al dialogo con l'opposizione. Avremmo voluto tuttavia un po' più di decisionismo e coerenza; infatti, qualcuno dovrà spiegare la *ratio* di smantellare la Sogin, ente ad alta tecnologia, disperdendo un patrimonio tecnico ed aumentando la disoccupazione. Nonostante queste nostre forti perplessità, dobbiamo pure riconoscere che alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento risultano condivisibili. Mi riferisco, in particolare alla lotta alla contraffazione ed alla tutela dei diritti di proprietà industriale, alle iniziative a favore dei consumatori in materia di trasparenza dei prezzi, alle reti o aggregazioni di imprese, all'ampliamento

su questo provvedimento non può essere positivo: anche se esso è stato migliorato con il contributo di tutti i Gruppi parlamentari, anche grazie all'accoglimento di alcuni dei nostri emendamenti, esso non risponde appieno alle urgenze e necessità sopra evidenziate. Non si fanno decisivi passi in avanti sul mercato dell'energia e del gas; si sprecano ulteriori occasioni per creare una reale concorrenza a vantaggio dei cittadini. Questo è un provvedimento che nel corso del suo lungo e complesso *iter* ha finito per diventare un calderone eterogeneo nel quale sono state inserite questioni per nulla o poco attinenti alla materia, in cui si ricorre allo strumento delle deleghe in bianco per problematiche che avrebbero piuttosto richiesto e meritato un maggiore approfondimento ed una più ampia discussione di quella finora svolta, in cui non si comprende come il Governo possa pretendere di mettere in campo ulteriori nuove iniziative, mantenendo

Signor Presidente, il Gruppo dell'IdV voterà no all'Atto Senato n. 1195, per molte buone ragioni che cercherò di illustrare nel tempo che mi è concesso. Mi riferisco innanzitutto all'*iter* che il provvedimento in esame ha avuto. Non possiamo infatti dimenticare le modalità con le quali il Governo e il relatore hanno stravolto il provvedimento in Commissione industria al Senato.

- emendamenti nuovi e riformulazioni di emendamenti già presentati, costringendo l'opposizione a presentare a sua volta subemendamenti. Tale meccanismo ha trascinato il provvedimento sino ad oggi in quest'Aula, raddoppiando di fatto gli articoli giunti dalla Camera. Soprattutto, non dimentichiamo che stiamo discutendo di un collegato alla legge finanziaria, quindi di un provvedimento funzionale alla realizzazione della manovra finanziaria, che dovrebbe attenere a settori di intervento precedentemente indicati nel DPEF e, oltre tutto, a contenuto omogeneo. Credo proprio che tutto si possa dire del provvedimento in discussione tranne che rispetti tali caratteristiche. Questo è il primo motivo di censura al provvedimento, che ci porta a dire e a votare convintamente no. Venendo al merito delle questioni, tratterò sostanzialmente, anche per motivi di tempo, la questione nucleare. Il ministro Scajola, nell'ottobre 2008, in una serie di interviste che aveva rilasciato, ha testualmente dichiarato: «Il Governo Berlusconi ha deciso il rilancio dell'opzione nucleare in Italia Al fine di creare un ambiente favorevole, il Governo sta procedendo all'istituzione della nuova agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, alla definizione dei criteri per l'individuazione dei siti nucleari e la qualificazione delle tecnologie,

se si crea un clima di fiducia nelle istituzioni e di trasparenza delle informazioni basata sulla capacità di governare le tecnologie necessarie». Pertanto, signor Ministro e colleghi della maggioranza, come pensate di creare un clima di fiducia e trasparenza avendo bocciato tutti quegli emendamenti, fra cui quelli dell'Italia dei Valori, che andavano in tale direzione? La vostra proposta politica - ci pare e ci occorre denunciarlo - va esattamente nella direzione contraria: volete una delega in bianco per scrivere nelle segrete stanze i decreti legislativi recanti i criteri per la disciplina della localizzazione degli impianti di produzione elettrica nucleare e dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi. forse per questo motivo che non avete voluto, come proponeva l'Italia dei Valori, che gli schemi legislativi avessero una seconda lettura da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Signor Ministro, colleghi della maggioranza, come pensate di facilitare l'accettazione delle tecnologie nucleari da parte delle popolazioni prevedendo la possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione, creando così una sorta di militarizzazione del territorio? Credo che in tal modo si vada nella direzione opposta. Anche non prevedendo la validità della autorizzazione unica all'ottemperanza della procedure di VIA e VAS, strumenti utili e necessari per conseguire complessivamente elevati livelli di tutela e qualità dell'ambiente, pare che si proceda nella direzione opposta. Quanto all'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, che ha il compito di garantire la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente, perché opporsi, come proponeva un emendamento del Gruppo Italia dei Valori, che l'Agenzia presentasse annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare, come fa qualsiasi *Authority*? rappresentanti del Governo, colleghi della maggioranza, noi crediamo che il deficit di modernizzazione, di innovazione e di efficienza nel mercato energetico del nostro Paese possa essere colmato solo integrando la politiche energetiche e climatiche in un contesto globale in cui sia assicurata la competitività economica e lo sviluppo sostenibile dell'ambiente. Invece, ci permettiamo di dire che con questo provvedimento il Governo sta facendo assumere al nostro Paese una posizione regressiva, fra l'altro indifferente alle indicazioni che arrivano dall'Europa. Come possiamo, infatti, signor Ministro, fare finta che non esista l'atto comunitario n. 32 sulla non proliferazione nucleare? In esso si evidenzia come negli ultimi anni il contesto politico ha indotto la comunità internazionale a concentrare la propria attenzione sulla riduzione dei rischi di proliferazione nucleare in sede di Nazioni Unite e G8, oltre che in altri ambiti internazionali. Nella sua comunicazione «Una politica energetica per l'Europa», la Commissione ha individuato la promozione della non proliferazione come una delle priorità fondamentali che devono essere perseguite per un'efficace politica esterna dell'Unione europea in materia di energia. La proposta politica dell'IdV andava, con gli emendamenti presentati, in una direzione opposta: era chiaramente antitetica rispetto a quella del Governo perché chiaramente volta all'attuazione e promozione di una strategia nazionale per lo sviluppo della filiera industriale nella realizzazione di tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e l'incentivazione della ricerca per la promozione delle tecnologie dell'efficienza energetica e per la loro integrazione. Per tali ragioni, l'Italia dei Valori aveva anche proposto la predisposizione di un piano operativo per la promozione della ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento al risparmio ed all'efficienza energetica, all'aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile, allo sviluppo, in particolare, del solare termodinamico ed al perfezionamento delle tecnologie per la cattura ed il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici.

la Lega Nord voterà a favore del provvedimento in esame. Il presente disegno di legge, collegato alla manovra finanziaria del 2009, anticipata il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è stato assegnato alla Commissione industria, successivamente allo stralcio di diversi articoli dal provvedimento originario, per le materie relative a sviluppo economico, competitività ed energia. Il provvedimento è stato adottato per affrontare alcune problematiche di natura strutturale che investono importanti settori strategici dell'economia del nostro Paese e che di fatto impediscono al nostro sistema produttivo di emergere da una situazione di generalizzato stallo economico. Gli argomenti all'inizio erano sostanzialmente riferibili a tre grandi aree di intervento, individuate nello sviluppo delle piccola impresa e dell'internazionalizzazione, nella tutela della proprietà industriale e della lotta alla contraffazione e nell'adozione di nuove strategie energetiche nazionali. rispondeva, infatti, alla necessità di approvare quanto prima il provvedimento in esame, proprio per la rilevanza strategica di alcune misure in esso contenute, le quali hanno l'obiettivo di ridisegnare la struttura del Paese, avviandolo verso una nuova fase di crescita e di sviluppo. I mesi sono, tuttavia, trascorsi e guardando al testo che oggi quest'Aula è chiamata ad approvare potremmo affermare che le cose non sono andate esattamente nella direzione indicata e, anzi, ci ritroviamo, oggi, un provvedimento molto più corposo rispetto al testo originario, nel quale durante l'*iter* in Commissione sono rientrati argomenti diversi che in qualche modo e in qualche caso hanno contribuito a creare qualche momento di confusione. Intendiamo, comunque, confermare la portata innovativa di alcune iniziative che rimangono fondamentali per spingere il Paese verso livelli maggiormente competitivi, anche alla luce dell'attuale fase di crisi economica e finanziaria. In questa ottica giudichiamo positive le misure che intervengono nel garantire lo sviluppo dell'apparato produttivo del Paese. Non dobbiamo dimenticare che le imprese, quelle piccole e medie imprese che caratterizzano le realtà locali dei nostri territori, rappresentano l'ossatura del sistema economico del Paese ed ogni azione volta a garantire la crescita delle stesse attraverso la creazione di sistemi di rete di piccole imprese, la promozione dei prodotti *made in Italy* sul mercato interno ed internazionale, il sostegno allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione deve essere necessariamente sostenuta a tutela delle piccole imprese del nostro Nord e, in generale, dell'apparato produttivo dell'intero

nonché il rifinanziamento degli interventi per la mobilità nelle fiere di rilievo nazionale. Riteniamo anche importante, in un'ottica federalista, l'approvazione dell'emendamento 11.305 che riconosce ai Comuni la possibilità di ottenere l'uso di un marchio comunale in relazione al proprio complesso patrimonio culturale, storico, architettonico ed ambientale ed anche per ciascun bene storico-artistico di relativa pertinenza. Saranno principalmente le imprese a raccogliere poi i frutti di quella azione politica intrapresa dal Governo in campo energetico che, di fatto, sancisce il ritorno dell'Italia al nucleare, il cui sviluppo, insieme alle altre fonti di energia alternative, non solo garantirà una minore dipendenza energetica verso altri Paesi, ma realizzerà anche una drastica riduzione dei costi dell'energia a vantaggio dell'intera collettività. La necessità di dare alle famiglie e alle imprese la possibilità di godere di un servizio elettrico efficiente e meno caro si concretizza anche all'interno di un nostro emendamento che è stato intervenendo in favore delle piccole gestioni esercenti servizi di pubblica utilità, si introduce un meccanismo graduale per l'applicazione delle sanzioni. Siamo certi di aver adottato misure che sono nell'interesse del Paese, come peraltro ci viene riconosciuto da diversi esponenti del mondo dell'imprenditoria e del lavoro. Ci ha fatto senz'altro piacere apprendere dal nostro Marco Loi, alla guida di una rappresentanza di lavoratori, che è stata evitata la chiusura dell'ALCOA di Portovesme, in Sardegna, salvando così il posto di lavoro ad alcune migliaia di operai. Siamo quindi felici di esserci presi in carico anche una problematica molto distante dalla Padania. Come dicevo, le risorse energetiche rappresentano un bene fondamentale per lo sviluppo e la ricchezza di ogni Paese, specie per un Paese come l'Italia, costretto all'assoluta dipendenza energetica nei confronti di altri. La soluzione al problema della differenziazione energetica e della sicurezza nell'approvvigionamento esiste e si chiama energia nucleare. Purtroppo non abbiamo alternative, dal momento che le stesse fonti rinnovabili da sole non riuscirebbero a soddisfare il nostro fabbisogno energetico, anche se ciò a cui dobbiamo puntare è lo sfruttamento di tutte le diverse fonti di energia disponibile. Il provvedimento ha quindi il merito di aver indicato la strada; tuttavia, dobbiamo avere il coraggio e la determinazione, ovviamente in sintonia con il territorio, di percorrerla fino in fondo. in fondo. Al riguardo esprimiamo soddisfazione per l'approvazione di una nostra proposta che circoscrive le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio nel settore energetico, introducendo elementi di maggior chiarezza e trasparenza. Alla luce di quanto detto, riteniamo che questo sia un provvedimento importante, di cui ringraziamo il Governo, il relatore, il Presidente e tutta la Commissione per il lungo ed articolato dibattito che ne ha accompagnato tutto l'*iter* di esame. Possiamo quindi ritenerci soddisfatti e dire ai nostri elettori di aver compiuto oggi un passo importante verso un futuro che sarà segnato da maggiore sviluppo e competitività.

determinando spesso anche elementi di contraddizione che sicuramente emergeranno nel corso dell'applicazione. Non rinunciamo però a mettere in evidenza alcuni elementi positivi contenuti nel provvedimento, segnalando l'apporto che dal Gruppo del Partito Democratico è stato offerto in spirito di servizio per mettere il Paese nella condizione di affrontare le emergenze che abbiamo di fronte. Abbiamo finalmente una qualificazione giuridica attendibile per le reti di imprese; abbiamo registrato l'impegno per garantire alle reti di imprese quegli strumenti di natura fiscale tali da assicurare le compensazioni interne e quindi costituire di per sé un fattore di incentivazione per le aggregazioni, tanto da restituire, quale elemento positivo, una nuova e diversa capacità competitiva delle stesse imprese; abbiamo registrato positivamente l'approvazione di alcune nostre proposte circa la semplificazione amministrativa e l'abolizione di pesanti, ridondanti e inutili procedure e certificazioni che per le imprese costituiscono un fattore di costo. A questo proposito, vogliamo augurarci che la clausola di salvaguardia approvata con l'articolo 33-*undecies* non vanifichi gli obiettivi e l'operatività contenuta in quegli articoli. quindi che quella norma di salvaguardia fosse posta a servizio della semplificazione e della snellezza dei procedimenti amministrativi. sottaciamo inoltre i passi avanti che è stato possibile compiere circa la tutela penale dei diritti di proprietà industriale e di contrasto alla contraffazione. Si sarebbe potuto fare di più, in una materia estremamente complessa, nella quale è necessario misurare gli strumenti perché gli obiettivi dichiarati possano essere

l'aver determinato una semplificazione nell'ordinamento giuridico e per gli oneri burocratici relativi alle società cooperative, in modo particolare quelle piccole. Detto questo, non possiamo non rilevare con forza alcuni fattori che temiamo possano produrre impatti molto negativi. Sono numerose le deleghe vaghe in qualche punto c'è una vaghezza che credo renderà vano anche il lavoro per la redazione di decreti legislativi immediatamente applicabili e coerenti con l'impianto comunitario. Al tempo stesso, verifichiamo, in modo particolare nel settore degli incentivi

e una certa contraddittorietà nelle norme d'immediata applicazione, sempre in tema di incentivazione per l'impresa. Troviamo poi non comprensibile la decisione così tenacemente sostenuta dalla maggioranza e dal Governo circa lo smantellamento di un patrimonio di conoscenze, oltre che di impresa ingegneristica, attraverso lo smembramento della Sogin e una decisione, che potrebbe risultare grave, circa il trasferimento non solo di quelle competenze e attività ma anche dell'attivo patrimoniale, in una materia estremamente complessa e delicata, quale quella dei siti contenenti rifiuti radioattivi o combustibili nucleari o sedi di dismesse attività nucleari, ad una società privata, a a patto che la stessa sia posseduta, per almeno il 20 per cento, da società a titolarità pubblica. Non ci sembra saggio inoltre depotenziare l'attività dell'ENEA non solo attraverso una trasformazione che metterà sicuramente nella condizione di nominare un nuovo organo amministrativo, obiettivo che normalmente può essere conseguito anche senza determinare smembramenti o smantellamenti di strutture operative quali l'ENEA,

nucleare attraverso il trasferimento di risorse umane e strumentali dall'ENEA e dall'ISPRA, depotenziando di fatto l'attività dell'ENEA, che riguarda non solo la sua funzione di agenzia del settore energetico, ma anche la sua funzione di accumulatore di saperi tecnologici che alimentano quei processi di trasferimento della conoscenza particolarmente utili a sostegno della piccola e media impresa. Ci appare rilevante la decisione assunta in ordine allo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi in terra ferma o in mare, che alimenterà quelle problematiche che sono state con forza segnalate dal presidente Zanda circa la subsidenza nell'area settentrionale dell'Adriatico

delle Regioni in ordine a materie particolarmente delicate, e definite dall'ordinamento costituzionale esattamente attraverso l'attribuzione di competenze in materia ambientale assegnata dall'articolo 117 alle Regioni, in una logica di concorrenza tra Regioni e Stato. determinato una modificazione della normativa nazionale, che di fatto espropria le Regioni in riferimento a quelle specifiche competenze, non significa, signor Ministro, aver eliminato ostacoli in relazione alla utilizzabilità dei giacimenti: ci accorgeremo che ciò significherà spesso crescita del conflitto e del contenzioso.

della salute dei cittadini ed a tutela dell'ambiente. Appare estremamente irragionevole la decisione di collocare in capo al TAR del Lazio la competenza, in maniera esclusiva per l'intero territorio nazionale, sui conflitti di natura ambientale in riferimento alle infrastrutture di natura energetica. Si sarebbe potuto fare di più sulle fonti rinnovabili, si sarebbe potuto fare di più per il risparmio energetico, attraverso la microcogenerazione, la generazione distribuita e la cogenerazione, per la quale esistono interventi positivi, seppur insoddisfacenti, alimentati dall'iniziativa del nostro Gruppo. Sul nucleare abbiamo detto parole molto precise, molto chiare, e riconfermiamo quella nostra preoccupazione. Vorremmo che si tornasse a discutere partendo dalle obiezioni che abbiamo formulato in quest'Aula e che non sono contestabili in alcuna misura. In conclusione, si alimenta un meccanismo che riporta il Paese indietro. Si rinuncia a liberalizzare il settore dell'energia e del gas, a riproporre i tetti *antitrust* per sostenere la nascita di un mercato in un settore particolarmente importante, nel quale registriamo registriamo un'assoluta dipendenza; si destruttura la difesa collettiva; si interviene sul sistema ferroviario e si smontano le riforme avviate per liberalizzare il nostro sistema produttivo e aprire il nostro sistema al mercato, alla concorrenza e alla competizione,

la nostra iniziativa non vuole e non vorrà mai rinunciare ad offrire un contributo per risolvere i gravi problemi che affliggono il Paese in questo momento.

ci accingiamo ad approvare un testo di importanza fondamentale, mi permetterei di dire storica, per i contenuti che rappresenta. In sostanza, una svolta radicale in tema di energia e un deciso scatto in avanti per quanto attiene allo sviluppo delle imprese. Lo dico, colleghi, con il duplice orgoglio in primo luogo di Presidente della Commissione industria, che tanto lavoro ed energie ha speso in questi ultimi mesi per giungere all'approvazione di questo provvedimento. A tal proposito mi sia consentito un doveroso ringraziamento al relatore, senatore Paravia, a tutti i colleghi della Commissione, per il prezioso apporto fornito al testo licenziato e, anche, un sentito ringraziamento ai colleghi dell'opposizione, in particolare al capogruppo in Commissione, senatore Bubbico, che pur nella diversità delle posizioni assunte, hanno comunque contribuito al raggiungimento di questo testo finale, oggi all'esame dell'Aula. secondo luogo, l'orgoglio è quello di membro di questa maggioranza parlamentare che, ancora una volta, ha mantenuto la promessa di voler metter mano, in senso costruttivo ovviamente, a temi ormai strategici per una nazione industrializzata quali, appunto, il riordino del sistema energetico e la previsione di misure concrete per lo sviluppo del settore produttivo. Non c'è Stato sociale, infatti, senza sviluppo e senza ricchezza nazionale. miliardi di euro all'anno: quattro punti di PIL, tanto è il costo della bolletta energetica che grava sulle famiglie italiane, ma soprattutto sui bilanci del sistema produttivo nazionale. Un onere troppo gravoso, che costringe il nostro il nostro tessuto imprenditoriale a difficili sforzi in termini di competitività, in particolare per le piccole e medie imprese che costituiscono la colonna vertebrale della nostra filiera produttiva. Ma non solo. Dipendere dal punto di vista energetico quasi interamente da altri Paesi condiziona non poco, da un punto di vista geopolitico, l'azione strategica dello sviluppo economico del Paese, rischiando addirittura la paralisi del sistema, come avvenuto qualche settimana fa con la vicenda della crisi tra i rapporti tra Mosca e Ucraina, dove le riserve di gas dell'ENI, che - ricordo - coprono il 54 per cento dei nostri consumi, sarebbero state sufficienti ancora per poche settimane, mettendo a serio rischio la sopravvivenza funzionale del Paese. A tal proposito, desidero ringraziare

La differenza tra il Governo attuale e quanto avvenuto in passato è l'assunzione di responsabilità tra chi vuole decidere e chi preferisce rimandare, cercando, con grave pregiudizio ideologico, di racimolare qualche voto da parte di qualche nostalgico ambientalista sopravvissuto. Il processo di avvicinamento alla produzione di energia da nucleare avverrà sotto comuni denominatori: sicurezza assoluta, rispetto per l'ambiente e garanzia della salute dei cittadini. Quindi nucleare sì, ma con tutti i presupposti di trasparenza e sicurezza necessari. Innanzitutto, la previsione di una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure; uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, di sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. È prevista, inoltre, la costituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare,

rilievo è 1'introduzione di misure a sostegno della creazione di reti di imprese e di promozione dello strumento degli accordi di programma, così come anche quelle tese ad incentivare il processo di internazionalizzazione del nostro sistema produttivo. cooperative, attraverso la creazione di un apposito albo delle imprese cooperative, e una serie di misure aventi come finalità la semplificazione delle procedure burocratiche tese al rilascio di titoli autorizzativi o concessori da parte della Importanti misure sono previste anche per la difesa dei diritti dei consumatori. Si parte dalla possibilità per l'utente di ottenere premi scontati in caso di sottoscrizione di polizze assicurative pluriennali, all'introduzione di importanti disposizioni a difesa della contraffazione e dell'originalità dei prodotti, azioni che combinate tra loro hanno tutte la stessa finalità: difesa di quel *made in Italy* che ci contraddistingue nel mondo per originalità e qualità dei nostri prodotti. Ma non basta. Anche grazie al lavoro svolto in Commissione industria attraverso l'indagine conoscitiva sui prezzi dei prodotti petroliferi al dettaglio, di cui sono particolarmente fiero per il contributo fornito all'abbassamento dei prezzi alla pompa, sono state introdotte nel provvedimento misure finalizzate alla conoscibilità dei prezzi dei carburanti, proprio per favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, mediante l'obbligo, verso chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante, di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato. È un segnale importante che denota l'impegno a tutela dei diritti dei cittadini contro il caro prezzo carburanti, a volte selvaggio, dovuto alle assurde oscillazioni del greggio sui mercati internazionali. Sempre in tema di sicurezza e a difesa della **Approvato** *(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)* 1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso alla infrastruttura La flessione della domanda di beni e servizi avrà un impatto occupazionale più evidente per le imprese industriali rispetto a quelle delle attività terziarie. Più contenuto dovrebbe essere il calo nel Nord-Ovest, mentre nelle altre Regioni si registrerebbe un calo pari al 2 per cento. Per questo è necessario intervenire, intervenire

È necessario incentivare le imprese, soprattutto quelle medio-piccole, dunque meno patrimonializzate, e garantire loro l'accesso al credito al fine di investire e mantenere i posti di lavoro. contenuto nell'attuale disegno di legge, che si vuole difendere con la forza di chi è convinto che presto possa tradursi in sviluppo e ricchezza per il nostro Paese. Il resto dipende da noi.

Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero rivolgere un ringraziamento sentito e non rituale ai membri della 10a Commissione, al suo presidente, senatore Cursi, al relatore, senatore Paravia, al vice ministro Urso, per l'attenzione, l'impegno e la sensibilità con cui hanno affrontato l'articolata e complessa materia oggetto del disegno di legge a breve, sarà sottoposto al voto finale di questa Aula. Il complesso dibattito in Commissione è stato caratterizzato da un confronto serrato, ma leale sulle questioni di merito. Anche le materie più delicate sono state affrontate in modo approfondito, con spirito costruttivo e fattivo. Un analogo clima si è sostanzialmente riprodotto nel corso della discussione in quest'Aula e di ciò ringrazio tutti i Gruppi, quelli di maggioranza per aver condiviso e sostenuto le proposte del Governo, quelli di opposizione per aver dimostrato senso di responsabilità raccogliendo, pur nella diversità delle posizioni, la nostra disponibilità costante al dialogo. Al di là delle questioni di metodo, il disegno di legge si segnala soprattutto per la rilevanza dei suoi contenuti. Il provvedimento interviene in un momento difficile contiene misure strutturali destinate a dare risposta concreta alle esigenze del sistema produttivo. Con questo provvedimento realizziamo riforme attese da anni, in grado di rilanciare la competitività del Paese e di promuovere lo sviluppo dell'economia reale. Con la disciplina delle reti di imprese puntiamo a contrastare la frammentazione del nostro tessuto imprenditoriale, offrendo alle aziende nuovi modelli di aggregazione che prescindono dai tradizionali vincoli territoriali. Dopo dieci anni di discussione finalmente il contratto di rete diventa legge e già si delineano le opportunità di crescita per le imprese che lo utilizzeranno. Anche il riordino degli interventi di reindustrializzazione e degli incentivi e delle agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione risponde ad una logica di razionalizzazione e di efficacia: le risorse non andranno più a programmi astratti e irrealistici, bensì a progetti mirati e concreti, con attenzione prioritaria al Mezzogiorno. Per sostenere e tutelare la nostra produzione all'estero abbiamo previsto la riforma degli strumenti di internazionalizzazione, il rafforzamento della lotta alla contraffazione e della tutela della proprietà industriale: sarà così possibile promuovere l'immagine del *made in Italy*. Un capitolo a parte è costituito dal pacchetto delle norme in materia di energia. L'insieme di queste misure è diretto a porre rimedio agli storici squilibri e ritardi del nostro Paese. Vorrei sapere se posso parlare.

al vostro posto, per cortesia.

il Senato non è in numero legale.

mi spiace dover protestare per la sua decisione

Grazie, Signor Presidente, l'Assemblea del Senato ha una sua dinamica, che può ben funzionare se i rapporti sono di fiducia, nei quali i Gruppi si sentono sempre tutelati. Noi oggi non ci siamo sentiti tutelati

Senatore Zanda, prendo atto del suo intervento. Le posso assicurare che in piena responsabilità ho assunto questa scelta anche perché ritenevo e ritengo che quando si fosse deciso all'unanimità di chiudere i lavori in serata, e quindi di andare avanti, vi fosse la volontà condivisa Grazie,

la invito a riflettere sulla complessiva gestione di questo argomento che ha visto, secondo me, una Presidenza che si è sforzata di essere quanto più imparziale possibile.

Presidente, la ringrazio per i chiarimenti. Vorrei però riportare la vicenda di questa sera all'interno di una normale dialettica parlamentare senza drammatizzare. Prendo atto, perché è nel suo diritto, che l'opposizione ha operato una scelta priva di *fair play*. È assolutamente all'interno dei suoi diritti regolamentari non partecipare al voto su un collegato senza avvertire la controparte, come

per ragioni tecniche, di una maggioranza e di un numero legale, che ovviamente ci sarebbe stato in termini normali, quando si ha l'appoggio da parte di almeno 12 colleghi dell'opposizione.

di aver fatto un tentativo, così come evidentemente da prassi era quasi naturale che fosse, ma non vorrei fosse drammatizzata una situazione nella quale le varie parti hanno giocato al limite di quella che è una normale dialettica parlamentare. Quindi la ringrazio, signor Presidente; parteciperemo con assoluta tranquillità a questa votazione e saremo qui domani, nel caso si dovesse confermare il risultato della precedente

la ringrazio, visto che avevo accettato stamani di poter intervenire a fine serata, comunque intervengo anche a quest'ora della notte. Intervengo per esprimere tutta la preoccupazione per una situazione molto grave che si sta per realizzare in Basilicata. Mi riferisco a dei cani, animali che se non si interviene urgentemente verranno deportati, come se fossero spazzatura. In Basilicata in questo momento si trovano in piccoli canili assistiti dal personale e da associazioni di volontariato. Ragioni meramente economiche hanno fatto indire delle gare di appalto, disertate da tutti perché la base dell'offerta era troppo bassa; di fatto, si è presentato soltanto un canile della Calabria: 3.000 posti per "accogliere" questi 420 cani. Mi sono appellata al Presidente della Regione, abbiamo oggi depositato un'interrogazione parlamentare e ci siamo rivolti

La legge sul randagismo stabiliva che i canili dovessero essere solo un malaugurato passaggio per un cane randagio, che poi avrebbe dovuto trovare una famiglia. Inoltre, le ASL di competenza dovevano condurre Con l'atto che sta per commettere la Regione Basilicata si cancellerebbero tutte queste leggi che nel corso degli anni l'Italia è riuscita a mettere in piedi. Mi auguro che il Senato se ne occupi e che non deleghi

quale senatore di montagna desidero ricordare con passione, riconoscenza ed affetto Achille Compagnoni, morto a 94 anni la notte scorsa, tra il 12 e il 13 maggio, all'ospedale di Aosta, dove era ricoverato da qualche giorno. Originario di Santa Caterina Valfurva, condusse vita militare per 18 anni, nel 5° reggimento alpini. Alpinista di buona fama, nel 1953 fu convocato da Ardito Desio per far parte della spedizione italiana che nel 1954 avrebbe tentato la salita al K2, la seconda montagna più alta del mondo. Superate le selezioni preliminari, Compagnoni partì per la spedizione, durante la quale ebbe funzione di braccio destro ed assistente del capo spedizione Ardito Desio. Il 31 luglio 1954, insieme a Lino Lacedelli (nato Cortina d'Ampezzo nel 1925), giunse sulla vetta del K2. In quell'occasione riportò il congelamento di alcune dita delle mani, che gli causarono un lungo ricovero al rientro dalla spedizione. Di ritorno dalla spedizione, Compagnoni ebbe a ridire con il Club Alpino Italiano per la proprietà delle riprese effettuate in vetta al K2, e successivamente utilizzate per il film «Italia K2», documentario ufficiale della spedizione. Negli anni successivi fu comunque molto attivo nel propagandare tale film presso scuole e sezioni CAI. Fu inoltre campione italiano di sci nordico e scalò il Cervino più volte per vie diverse. Compagnoni era guida alpina a Valtournanche e faceva l'albergatore a Cervinia. Ricordiamo anche che nel 1955 gli fu data la medaglia d'oro al valor civile per «il luminoso esempio delle più alte virtù di nostra gente». A lui, un uomo della montagna, un sentito e doveroso pensiero di ringraziamento per aver onorato la montagna e la gente di montagna e per il lustro che vi ha dato. Fa inoltre piacere ed è doveroso in questa Aula ricordare un normale e semplice cittadino. Ai familiari ed amici le più sentite condoglianze ed un forte abbraccio. Signor Presidente, intervengo per sollecitare il Governo al rispetto di un impegno assunto, in particolare dal sottosegretario Vegas, con l'ordine del giorno G3.124, in sede di finanziaria, e con il successivo ordine del giorno G11.0.700, in sede di esame del disegno In sostanza, con tale ordine del giorno si impegnava il Governo a chiarire, entro il 30 aprile 2009, attraverso un'interpretazione autentica, limitatamente ai soggetti ricompresi nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, che nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge, avesse interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al dicembre 2002, lo stesso non sarebbe stato tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS. L'urgenza, signor Presidente, così come avevo già Grazie,

550 e 918, finalizzato al riconoscimento della sordocecità come disabilità unica e specifica, sulla base degli indirizzi contenuti nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche, approvata il 12 aprile 2004